L'ordine del giorno reca: «Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri». Ricordo che nella seduta di ieri, al termine della discussione sulle sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, del senatore Gasparri ed altri, e n. 2, della senatrice Finocchiaro ed altri. Intervenendo in replica alla discussione, l'onorevole Berlusconi ha posto a nome del Governo la questione di fiducia sull'approvazione della proposta di risoluzione n. 1.

È in arrivo.

ad un vergognoso teatrino della politica, che ha fatto male alla credibilità delle istituzioni e all'azione del Governo e soprattutto ha lasciato disorientati i cittadini e gli elettori che credevano, con il loro voto, di avere dato una chiara indicazione su chi dovesse governare il Paese per l'intera legislatura. La Lega Nord non ha mai partecipato a questa farsa: abbiamo sempre cercato di abbassare i toni e abbiamo cercato di ricucire con tutti, nel modo più responsabile possibile, senza però mai dimenticare il patto stretto con i nostri elettori. Dall'inizio della legislatura siamo stati i più presenti in Parlamento. Non abbiamo mai fatto mancare il sostegno al Governo. Siamo sempre stati leali. Nel nostro Gruppo non vi è stato alcun tentennamento, nessun cambio di casacca. Siamo sempre stati uniti, compatti e granitici agli ordini di Umberto Bossi. Lo abbiamo fatto convinti che, prima di tutto, viene il rispetto per i nostri militanti che attaccano i manifesti, che distribuiscono i volantini, che organizzano gli incontri pubblici e i gazebo nelle piazze; i nostri elettori, che non ci hanno eletto per partecipare al teatrino della politica, o per fare continue ed inutili polemiche: ci hanno eletto solo ed esclusivamente per dare risposte alla nostra gente, al nostro

Siamo riusciti a realizzare riforme importanti e, grazie al ministro Bossi, abbiamo quasi concluso il percorso del federalismo fiscale. Poi è arrivato lo strappo dei finiani, con la costituzione dei Gruppi parlamentari, che ha iniziato a logorare l'azione del Governo, creando polemiche e scontri politici. I primi a lamentarsene sono stati i cittadini, che non ne hanno capito le ragioni. Negli ultimi sei mesi c'è stata una *escalation* di dichiarazioni e di comportamenti che ai più sono apparsi incomprensibili. Il 28 luglio Fini dichiarava: «Insieme a Berlusconi per onorare l'impegno politico». Il 3 agosto sempre Fini dichiarava: «Il terzo polo non è la mia idea. Noi leali al Governo». A settembre i finiani hanno votato la fiducia, ma da lì in poi non hanno perso occasione per attaccare sistematicamente il Governo, fino ad arrivare alle creazione dell'ennesimo nuovo partito, alla nascita del cosiddetto terzo polo e, infine, alla presentazione della mozione di sfiducia alla Camera, l'errore più grave che hanno commesso. Per quanto ci riguarda, troppe contraddizioni, troppe dichiarazioni avventate, troppi cambi di rotta. Colleghi di Futuro e Libertà, in politica contano coerenza e credibilità, e voi avete dimostrato di non avere né l'una né l'altra. Questa è la realtà, e i cittadini lo hanno già capito. In questi mesi abbiamo sentito Fini annunciare l'intenzione di fondare un nuovo centrodestra moderato, alternativo a quello attuale. La cosa che non regge e che i cittadini non capiscono è come sia possibile fondare un centrodestra moderno con Casini, che è un vecchio democristiano e che solo la settimana scorsa ha dichiarato che si stava meglio nella Prima Repubblica, e con Rutelli, che è stato candidato Premier per il centrosinistra e cofondatore del Partito Democratico. E, soprattutto, la gente si chiede: come mai, per 15 anni, avete sempre sostenuto Berlusconi senza mai criticarlo? Come mai per 15 anni Berlusconi vi è sempre andato bene? Forse perché l'alleanza con lui vi ha permesso di conquistare poltrone, posti in Parlamento, di Governo, nelle Regioni e negli enti Questo è quello che pensano i cittadini. Oggi vedremo quanti eletti nel centrodestra parteciperanno al tentativo di ribaltone voluto da Fini e dal centrosinistra. Perché è giusto ricordare anche questo: siamo l'unico Paese al mondo dove le opposizioni, che hanno perso le elezioni, in un momento di crisi della maggioranza non chiedono il voto, ma si muovono per ottenere posti in un cosiddetto Governo tecnico È evidente a tutti che non vogliono il voto per una ragione sola: hanno paura, sanno bene che i cittadini non si sono dimenticati i danni e i disastri che hanno fatto quando loro erano al Governo *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Hanno paura di perdere, per l'ennesima volta, le elezioni. Ma noi su questo vogliamo essere molto chiari. Non permetteremo mai un Governo dei perdenti. Dovete mettervelo bene in testa, cari colleghi dell'opposizione. In questo Paese governa chi vince le elezioni. Voi le avete perse e non avete alcun diritto di governare. voglio aprire una parentesi, cari colleghi del centrosinistra. Smettetela. Smettetela di cavalcare in modo demagogico la protesta degli studenti. La riforma dell'università che stiamo per approvare poteva forse avere più risorse: per ora abbiamo stanziato 1 miliardo di euro, che in questo momento di crisi non è poco. Inoltre, abbiamo inserito incentivi che andranno a premiare gli atenei virtuosi, senza penalizzare gli studenti. In Inghilterra, i giovani stanno protestando perché hanno aumentato le rette universitarie a 9000 sterline all'anno, ovvero 1000 euro al mese.

e condannate senza "se" e senza "ma" i violenti dei centri sociali che anche oggi sono alla testa dei cortei nelle piazze; centri sociali che avete sempre aiutato e finanziato. Questo bisogna sempre ricordarlo. Ciò detto, non dobbiamo nasconderci che i problemi politici di oggi sono collegati anche al fatto che questo Governo ha intrapreso un percorso di riforme con l'obiettivo di cambiare il Paese e che c'è qualcuno, anche fuori dal Parlamento, che queste riforme non le vuole. Il federalismo fiscale, le riforme istituzionali, la fine del centralismo e dell'assistenzialismo sono il terrore di chi non vuole il cambiamento. I Palazzi romani, i poteri forti, le varie cricche di Stato stanno reagendo: non vogliono perdere il loro potere e sono i primi in questo momento a sostenere chi crea instabilità. Hanno giornali, uomini, i "Montezemoli" di turno, pronti a muoversi. Sono quelli che, pubblicamente o sottobanco, auspicano la nascita di nuovi Governi tecnici. E per chi non l'avesse ancora capito, i Governi tecnici servono a una cosa sola: a bloccare le riforme e il cambiamento in questo Paese. Governo).* In conclusione, invito tutti gli eletti nella maggioranza a riflettere, ad abbandonare i personalismi, a smetterla con l'ipocrisia e a pensare solo al bene del Paese. Lo dico soprattutto ai colleghi di Futuro e Libertà Le critiche costruttive vanno sempre bene, ma è stando all'interno della maggioranza che si può costruire qualcosa di positivo. Abbandonare la maggioranza per schierarsi con la sinistra ha un solo significato: tradire il mandato elettorale. Pensateci bene prima di farlo. Oggi e nei prossimi giorni ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. La Lega Nord vuole continuare a governare. Il nostro obiettivo, però, presidente Berlusconi, non è arrivare a fine legislatura e basta. Il nostro obiettivo è arrivare a fine legislatura cambiando il Paese e realizzando finalmente le riforme. Se avremo i numeri per farlo andremo avanti con l'azione di governo, altrimenti - lo abbiamo già detto in diverse occasioni - l'unica strada possibile è il voto. La Lega, presidente Berlusconi, non cambia idea e le rinnova convintamente la fiducia.

signor Presidente del Consiglio, il voto di fiducia di oggi non è semplicemente il trentottesimo che il suo Governo chiede al Parlamento dall'inizio di questa legislatura. È il voto che, tra il Senato e la Camera, sancisce la conclusione di un'epoca politica. Il diniego della fiducia da parte della seconda componente della sua maggioranza, guidata da Fini, chiude la stagione iniziata 17 anni fa, quando lei si impegnò in politica dichiarandosi in favore proprio di Fini nella sfida che allora ci contrapponeva per la elezione a sindaco di Roma. Lei ha già perduto il sostegno della componente centrista e cattolica guidata da Casini;

Sono proprio i moderati, dunque, a chiedere di concludere questa esperienza di Governo. Alleanza per l'Italia è nata per contribuire all'uscita dal fallimento di questo bipolarismo guerriero, che si è arenato ormai sulle posizioni dominanti, come abbiamo sentito, non certo dei moderati, ma delle forze estreme, e che ha permesso, tre volte al centrodestra e due al centrosinistra, di vincere le elezioni,

e si capisce bene che tutti gli annunci rinnovati ieri - dal piano mirabolante per il Sud, al prodigioso federalismo a beneficio del Nord, dalle riforme della giustizia fino alla liberazione dai rifiuti nel napoletano - sono invenzioni. Non avete avuto la forza di realizzarli con la più grande maggioranza della storia della Repubblica, non ce la farete certo sul filo di un paio di voti. Quello che le abbiamo proposto con la convergenza del nascente polo formato da ApI, UDC, FLI, MpA e dalle altre componenti democratiche, moderate e riformiste è di prenderne atto e di creare le condizioni per una larga maggioranza di forze responsabili.

coraggiose, le riforme necessarie capaci di riportare l'Italia sul terreno della crescita, del lavoro e della competitività; di garantire stabilità, ripristinando l'avanzo primario per i conti pubblici. Ma lei ha detto no; per quasi tre anni, no alle riforme, («non si fanno in tempi di crisi» ha detto Tremonti): liberalizzazioni, fisco, mercato interno europeo, *green* *economy*, giustizia civile, famiglia. Da tre anni, no a risparmi e tagli di bilancio che non fossero assurdamente lineari, mentre la Germania ne ha operati di più severi dei nostri, ma ha accresciuto gli investimenti in ricerca, università, scuola, formazione, cultura. Da quando la crisi è esplosa, no a serie misure anticorruzione; no al taglio dei costi della politica, che noi di ApI abbiamo proposto più e più volte in Parlamento. Oggi, lei dice no a un nuovo Governo di ampia responsabilità nazionale, capace di affrontare queste scelte difficili. Si arrocca. Ma non si sorprenda se milioni di elettori moderati guarderanno con sempre maggiore interesse al nuovo polo che viene formandosi, con l'incontro di forze e personalità provenienti da diversi schieramenti. Perché è il tempo di unire, non di dividere ancora, e su orizzonti sempre più ristretti. Di governare, non solo di polemizzare contro gli avversari. Di rendere alle istituzioni i compiti alti che la Costituzione assegna loro: un Governo forte; un Parlamento libero; istituzioni di garanzia e controllo degne e solide; poteri locali e regionali più efficienti, vicini ai cittadini, parte decisiva dell'unità nazionale. Per questo confidiamo, con il nostro voto contrario, che per una maggioranza che finisce, per un Governo che passa la mano, si creino le condizioni di una nuova, ampia maggioranza, urgentemente al lavoro per il bene dell'Italia. Ci rifletta, signor Presidente del Consiglio. Non illuda nessuno che il ricorso a elezioni anticipate possa risolvere - con maggioranze più piccole, con consensi più ridotti - ciò che non si è risolto finora. Faccia subito, dopo il voto del Senato, il passo che la restituirebbe alla considerazione di tutti gli italiani. Non più l'uomo di parte che non ce l'ha fatta, ma l'uomo della Repubblica che si pone, nel momento più difficile, al servizio di tutto il popolo italiano. *(Applausi Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, onorevoli colleghi, mi consentirete innanzitutto di iniziare il mio intervento con una riflessione rispetto alle considerazioni che mi ha rivolto, e ci ha rivolto, il capogruppo della Lega, senatore Bricolo. Senatore Bricolo, cercherò di dimostrare, con il mio intervento, che abbiamo a cuore, almeno quanto lei, il rispetto del patto con gli elettori e la consapevolezza che quando si costruisce un'alternativa politica, quell'alternativa passa inevitabilmente attraverso il consenso popolare. rivolgo al senatore Bricolo, perché appartengo ad una storia politica che non ha la cultura del ribaltonismo. Vorrei ricordare al senatore Bricolo che noi non siamo mai stati ribaltonisti, né ieri, come è capitato come è capitato ad altri, né oggi, né domani.*(Applausi dal Gruppo FLI).* Piuttosto, vorrei invitare il senatore Bricolo, per coerenza rispetto alla sua riflessione, ad evitare di essere complice di un ribaltone. Perché, caro senatore Bricolo, la maggioranza che ha vinto le elezioni - come le ha ricordato stamattina un illustre commentatore è la maggioranza che aveva non solo la *leadership* consolidata, forte, responsabile di Umberto Bossi, ma aveva una diarchia di *leadership* all'interno del centrodestra. Il centrodestra che si è presentato agli elettori non era un partito, era una lista, quella del PdL, dove confluivano più storie politiche, tutte con pari

a chi non ha la memoria lunga della storia politica italiana - che proprio quella diarchia di *leadership* aveva determinato, o contribuito a determinare, il successo del centrodestra: quel centrodestra che, anche grazie a quel contributo, aveva ottenuto quel premio di maggioranza che consente di governare e di garantire - almeno sulla carta, almeno sul dato quantitativo - la stabilità di governo.

peccato che non abbia ricordato il giorno dopo, il 29 luglio, quando, nonostante le considerazioni alle quali lei faceva riferimento, l'ufficio politico del PdL ha ritenuto di dichiarare incompatibile con il PdL stesso il cofondatore del partito, onorevole Gianfranco Fini, determinando un processo politico che ha come causa fondamentale quella che io definisco la pretesa dell'autosufficienza. che ha dato luogo ad un enorme errore politico, rispetto al quale ancora oggi rischiamo di pagare le conseguenze. Lo dico, senatore Bricolo, perché se si rompe quel patto, se si determina quella rottura, non c'è altra strada rispetto alla crisi. In altri termini, la risposta è duplice: o la ricomposizione del centrodestra, che è l'unico elemento di recupero di coerenza e di rispetto sostanziale del patto elettorale, oppure un'altra maggioranza, quindi il ribaltone,

che sono stati eletti all'opposizione, che sono stati eletti nell'UDC, che sono stati eletti nell'IdV, che sono stati eletti in altre forze politiche e partitiche. Attraverso un'operazione legittima - come la vogliamo chiamare? di trasformismo e di transumanza parlamentare, determino eventualmente una maggioranza alla Camera dei deputati, che sarà in grado - forse di fare aritmetica parlamentare, ma non di determinare le condizioni per uscire dal tunnel della crisi e garantire la stabilità. Rispetto a questo bivio, vale a dire o la ricomposizione del centrodestra o il ribaltone di stabilità, noi ci permettiamo, signor Presidente del Consiglio, di fare un'altra proposta,

- sarà solo per un eventuale nuovo Governo di centrodestra; e se il Presidente del Consiglio dovesse ricevere la fiducia alla Camera, non c'è altro spazio che per un ruolo di responsabilità. Noi riteniamo però, signor Presidente del Consiglio,

nella nostra storia politica, con il consenso popolare. Vorremmo che il consenso popolare fosse pieno attraverso una nuova legge elettorale

credo che ci sia un'alternativa a questo bivio e che questo passi attraverso un percorso di comune e chiara responsabilità politico-istituzionale. Signor Presidente del Consiglio, il ruolo più significativo ed importante ce l'ha lei, perché se lei va alla Camera e va alla conta parlamentare segnala tre sconfitte, non una vittoria. Primo, la sconfitta della *leadership*, perché la capacità della *leadership* è capacità di costruire un punto di sintesi e di compromesso alto. Questa è la politica. Secondo, lei rischia di fatto il ribaltone. Terzo, lei rischia di fatto di determinare l'instabilità di governo. Signor Presidente del Consiglio, con chiarezza di posizioni... Presidente, io so distinguere tra la politica e i gazebisti, cioè i professionisti del gazebo e della propaganda. *(Commenti dal Gruppo LNP).* Chiuso questo inciso, per rivolgermi ancora al Presidente del Consiglio,

Signor Presidente del Consiglio, le propongo questo percorso politico-parlamentare. Le chiedo, rispetto al dibattito che si sta svolgendo in quest'Aula, rispetto al dibattito che si è svolto e si svolgerà alla Camera, di prendere atto delle risultanze del dibattito. Il Senato voterà, presumibilmente dando la fiducia dando la fiducia al Governo. Rispetto alla fiducia al Governo io le chiedo, il momento dopo, di prendere atto di questa fiducia, di recarsi al Quirinale, di aprire...

Signor Presidente del Consiglio, per accompagnare questa proposta e per concludere questa immagine, noi, rispetto alla richiesta di fiducia, voteremo con l'astensione, per accompagnare questo processo. Per accompagnare questo processo, noi voteremo con l'astensione. E mi consenta, signor Presidente del Consiglio, al di là del fastidio*... Colleghi, il senatore Viespoli sta per terminare il suo intervento.

Colleghi, chi non è interessato può uscire dall'Aula: c'è troppo chiacchiericcio. Sospendo la seduta, eventualmente. *(Brusìo).* Non si può lavorare così. Mi costringete a sospendere la seduta, colleghi: è la seconda volta che lo dico.

Colleghi, guardate che sto per sospendere la seduta. Per cortesia, i signori Capigruppo sono invitati a fare in modo che i loro colleghi stiano in silenzio. Senatore Belisario, inizi.

Presidente, io ho buona volontà, però vorrei che anche i colleghi, il Governo e il Presidente del Consiglio avessero la pazienza di ascoltare. Probabilmente dirò cose che la maggioranza e il Presidente del Consiglio non gradiranno, ma la regola del Parlamento è di ascoltare, come noi abbiamo ascoltato e ascolteremo, senza disturbare. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, poco più di due mesi fa lei, signor Presidente del Consiglio, è venuto in quest'Aula per chiedere la fiducia. L'Italia dei Valori cercò di spiegarle, e pensava di essere stata chiara, che per il bene del Paese fosse giunto il momento che lei abbandonasse il *bunker* di palazzo Chigi, passasse la mano, dichiarasse il fallimento della sua azione politica. Sono passate solo poche settimane e ritorna qui, ancora una volta, con la consueta faccia di bronzo - mi perdoni - a richiedere la fiducia. È evidente che ella è sprezzante della sacralità del Parlamento e del popolo italiano; ritiene che tutto sia una favola, anche la vita e le sofferenze di questo Paese e degli italiani, che invece sono reali. Ma Presidente, siccome la pazienza c'è, poi dirò qualcosa, perché *repetita iuvant*. Vediamo se riusciremo ad essere più chiari:

I mezzi di informazione e di comunicazione, specie quelli pubblici e privati televisivi, che lei controlla nella maniera più militare possibile, descrivono la città di Roma, la nostra capitale, come una città blindata. Addirittura vi sarebbe una zona rossa in cui migliaia di uomini presidiano il Parlamento. Ma, Presidente,

una democrazia normale che noi dobbiamo far valere nella dialettica, nella polemica, nel contrasto duro, ma nella civiltà di poter tutti esprimere fino in fondo le nostre opinioni. Lei, Presidente, parafrasando Cicerone, sta abusando della pazienza del Parlamento e degli italiani. degli italiani. Lei, Presidente del Consiglio, è ormai sfiduciato da un Paese in sciopero generale contro la sua politica, che affama, degrada, corrompe la nostra società. Studenti e docenti, magistrati ed avvocati, imprenditori e lavoratori, giornalisti, precari, forze dell'ordine, terremotati, famiglie sempre più povere sono in grande e straordinaria agitazione. Parlano alle coscienze di tutti noi e dovrebbero parlare alla sua coscienza (se, come spero, lei conserva una coscienza). Lei è il più incredibile Presidente del Consiglio che sia esistito. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Si prega di controllare il Devoto Oli, e probabilmente ne capirete il senso. ha sempre pensato che l'Italia sia come un'azienda, una delle sue aziende, ma l'Italia, Presidente, è una Nazione straordinaria che si governa con le azioni concrete, che si ama, e non si compra. Già, comprare! Un verbo usato in questi giorni: lei è il mandante politico della più grossa compravendita di parlamentari!

Io la invito a fare il Presidente del Senato.

deprecabili e condannabili sempre, perché sono in odio agli elettori, oggi sono favoriti dal suo *entourage* solo per fornirle qualche voto in più per sopravvivere a se stesso. Non è nuova la mia espressione. Ma in presenza di una maggioranza sbriciolata nei fatti anche il dibattito dei giorni scorsi, dalle ultime ore, di questa mattina, lo va confermando ha spiegato agli italiani a cosa serve l'accanimento terapeutico usato per tenere in vita un Governo che ha l'elettroencefalogramma ormai piatto da mesi? e LNP).* Lei sa benissimo che nel momento in cui mette fuori il piede da Palazzo Chigi dovrebbe essere accompagnato al tribunale di Milano per subire il processo che - lei lo sa - ha un esito già segnato, perché, se i magheggi legislativi del suo Ministro della giustizia non lo avessero già impedito,

Vede, Presidente del Consiglio, lei vuole bene solo a se stesso: e non importa se questo Paese va in malora, non importa nemmeno se le diplomazie che contano non si fidano più di noi e del suo colossale, incredibile conflitto d'interessi. Per questo, lei se ne deve andare: per restituire al Paese la serenità che continua a togliergli, il sorriso alle famiglie ormai senza speranza, il futuro ai giovani che vivono nell'incertezza. E poi, la smetta di dire che i conti pubblici sono in ordine... E poi, la smetta di dire che i conti pubblici sono in ordine, che non ha messo le mani nelle tasche degli italiani, che la spesa pubblica è diminuita: lei sa bene che così non è. Lo sa anche il Ministro dell'economia, lo dimostrano i dati pubblicati, conosciuti ed elaborati da studiosi ed economisti (sono i dati dell'ISTAT, di EUROSTAT): negli anni in cui lei ha governato, il debito pubblico è aumentato di 490 miliardi di euro. Le cifre sono pubblicate, non sono una mia invenzione né un'invenzione dell'Italia dei Valori: parliamo di 8.000 euro a testa

hanno portato la pressione fiscale dal 45,4 al 47,2 per cento. La spesa pubblica - lo sa bene, ce lo dice la Corte dei conti - è ormai fuori controllo. se noi siamo in queste condizioni, se il Paese è in queste condizioni, lei faccia un atto di resipiscenza operosa. Vada al Quirinale, rassegni le dimissioni e dica al Paese: ci ho provato, ho fallito, me ne vado*. Signor Presidente, ieri abbiamo ascoltato con estrema attenzione, come era nostro dovere, gli argomenti che lei ha formulato qui al Senato per motivare la sua richiesta di un nuovo voto di fiducia, rivendicando le azioni compiute dal suo Governo, soprattutto in materia di politica economica, oltre alla solita enunciazione di ambiziosi e futuribili progetti di riforma, che costituiscono il canovaccio tradizionale del suo programma politico. Abbiamo anche preso atto di questo richiamo alla responsabilità e alla lealtà che lei ha rivolto ai parlamentari, oggi di FLI eletti nelle liste del PdL, quasi evocandone una sorta di crisi di coscienza personale. Abbiamo anche preso atto che lei non ha rivolto alcun invito ai parlamentari del MPA, malgrado noi siamo stati eletti con la nostra lista nel 2008 all'interno di una coalizione da lei guidata, perché ben consapevole di non poter richiamare il Movimento per le Autonomie ad una pretesa lealtà nei confronti dell'Esecutivo, perché sa bene chi tra noi ha disatteso i patti. Noi abbiamo stipulato nel 2008 un'alleanza politico-elettorale con la coalizione da lei guidata sulla base di un accordo preciso, che non si fondava su schematismi politico-ideologici, che non ci interessano, né sui modelli tradizionali di questo bipolarismo muscolare italiano, ma trovava fondamento, in coerenza con la nostra ragione costituiva - quella di tutelare l'interesse di un territorio, da vero movimento autonomista - in un accordo che aveva come oggetto unico ed essenziale lo sviluppo del Mezzogiorno. È in questo che lei ed il suo Governo avete mancato al patto. Abbiamo dovuto registrare in questi 31 mesi un totale disimpegno dell'Esecutivo dalla responsabilità che aveva assunto di fronte agli elettori meridionali. Per lei, il Mezzogiorno è soltanto *marketing* politico, è soltanto *spot* elettorale cui non rivolge alcuna reale attenzione, perché la sua cultura politica, il suo radicamento sociale, le sue relazioni privilegiate sono tutte dentro l'area forte del Paese, il Nord. La presenza in modo così decisivo di un partito come la Lega, che interpreta correttamente la propria parte, ha determinato lo spostamento oggettivo del baricentro degli interessi del Governo nella direzione delle aree più ricche del Paese. In questo senso, signor Presidente, è emblematico quello che è accaduto con il tema del Fondo per le aree sottoutilizzate, che non è un tormentone insopportabile volto ad infastidirvi, ma si tratta della scelta strategica di politica economica attraverso cui avete operato in questi anni, in questa fase congiunturale. Voi avete sottratto le risorse del Mezzogiorno per gestire la crisi economica italiana. In un confronto del tutto informale, qualche giorno fa, il vice ministro Castelli mi diceva, con grande sincerità: «Attraverso i fondi FAS abbiamo salvato l'Italia». lo non credo che voi abbiate salvato l'Italia: di certo, avete garantito il mantenimento di livelli di benessere delle aree più ricche del Pese, impoverendo il Sud e sottraendogli le risorse destinate a colmare il divario che si è, invece, ulteriormente allargato. Una sorta di Robin Hood alla rovescia, signor Presidente: ha tolto ai poveri per dare ai ricchi! Durante il dibattito sulla scorsa fiducia a settembre, lei, signor Presidente, mi fece pervenire un biglietto con il quale, in qualche modo, mi contestava il mancato utilizzo delle risorse del FAS per il periodo di programmazione 2000-2006 da parte delle Regioni meridionali. Il suggeritore interessato di quella nota, il ministro Fitto, oltre a trarla in errore, dimostrandosi inopportuno e inaffidabile, le ha dato un'informazione faziosa, come del resto è sempre stata l'azione del Ministro in questa vicenda. Il ministro Fitto le ha taciuto, per esempio, che il mancato utilizzo di quelle risorse è in gran parte addebitabile alle grandi agenzie di spesa nazionale, l'ANAS e le Ferrovie dello Stato. I fondi trasferiti dalle Regioni, cioè soldi delle Regioni, attraverso accordi di programma quadro, da queste grandi agenzie di spesa sono stati utilizzati, secondo gli ultimi dati, soltanto per un ammontare pari all'8 L'ANAS, per esempio, in Sicilia, dei 2,2 miliardi di euro trasferiti ha speso in 10 anni solo 150 milioni di euro. Chieda conto di questo all'ANAS invece di affidarle, attraverso un commissariamento illegittimo, la gestione delle autostrade siciliane. Voi ritenete di affermare il principio che, di fronte ad un Mezzogiorno incapace di spendere in modo efficiente, la logica è quella di requisire le risorse destinate al suo sviluppo attraverso una gestione centralistica che si nutre di poteri vessatori e sostitutivi. È questo l'assioma che presiede ed assiste tutto il Piano del Sud. Signor Presidente, avremo un Paese in cui, mentre al Nord si riconosce una prospettiva di federalismo avanzato e di forte responsabilità territoriale, al Mezzogiorno questo stesso titolo viene negato, perché se ne dichiara una sorta di subalternità culturale e di minorità genetica, per cui noi non siamo nelle condizioni di affrontare questa sfida della responsabilità. Signor Presidente, noi allora non ci fidiamo. Abbiamo avuto prove conclamate che il patto politico sancito con il Movimento per le Autonomie lei non l'ha rispettato; ma, cosa ancor più grave, non ha rispettato il patto morale che ha stipulato con gli elettori meridionali. Lei, quando vuole enfatizzare il suo impegno per il Mezzogiorno, non sa andare oltre il richiamo alla sua azione per rimuovere l'immondizia dalle strade di Napoli. Non mi sembra che l'immondizia sia stata rimossa e, comunque, questo non mi pare certo un gran titolo per meritare la fiducia dei meridionali. Signor Presidente del Consiglio, il Sud ha bisogno di un interlocutore più affidabile e, probabilmente, il Paese ha bisogno di voltare pagina. Per questo, non voteremo la fiducia. Signor Presidente del Consiglio, l'Unione di Centro le negherà la fiducia come ha già fatto per 37 volte dall'inizio della legislatura. Non è una questione di principio, né uno sterile capriccio da oppositori, ma un atto di lealtà e di trasparenza nei confronti dei nostri elettori che vogliono qualcosa di più e di diverso dal Governo di un Paese importante come l'Italia. Dunque, quello che esprimeremo è un no responsabile in favore degli italiani, quindi, e non una manovra di palazzo con cui cercate di liquidare questo delicato e importante passaggio parlamentare. L'Unione di Centro ha dimostrato con i fatti la sua coerenza, essendo stata all'opposizione di Prodi ieri e del suo Governo oggi, e lo ha fatto sottoponendosi sempre e senza paura o reticenza al giudizio degli elettori. Siamo l'unica forza moderata presente in Parlamento a non essere stata costretta a fare alleanze anomale, come quelle che lei da un lato ed il Partito Democratico dall'altro avete fatto alle ultime elezioni, consegnando il bastone di comando del Governo alla Lega e quello dell'opposizione prima a Di Pietro e oggi anche a Grillo e a Vendola. Per questo, non accettiamo lezioni di coerenza, di lealtà e di trasparenza. E proprio perché siamo consapevoli delle nostre buone ragioni, abbiamo il dovere di parlare il linguaggio della verità in Parlamento e nel Paese. La verità, signor Presidente, è che questo sistema politico non funziona perché non garantisce né l'efficienza del Governo, né l'efficienza del Parlamento: del Governo, perché espressione di un sistema elettorale falsamente bipolare con cui si formano solo alleanze elettorali incapaci di governare il Paese (è successo a Prodi nei due anni del suo Esecutivo triste, sta accadendo a lei che due anni e mezzo fa aveva 100 parlamentari in più a sostegno del suo Gabinetto, ed oggi si trova senza maggioranza politica e forse numerica); del Parlamento, unica e vera sede della sovranità popolare come dice l'articolo 1 della Costituzione, i cui membri purtroppo sono nominati, e non scelti dagli elettori, elettori, con un premio di maggioranza che trasforma una minoranza organizzata in una vasta maggioranza parlamentare al cui arbitrio sono affidate scelte importanti e strategiche per tutto il Paese. Per questi motivi, signor Presidente del Consiglio, ci saremmo aspettati da lei un intervento chiaro e netto sui limiti di questo sistema che non garantisce il bene dell'Italia imprigionandola nel populismo, nella contrapposizione frontale di tutti contro tutti, nella logica feroce del «tanto peggio tanto meglio». Da lei, signor Presidente, che tanti anni fa ha saputo interpretare le esigenze di cambiamento della politica italiana, ci saremmo aspettati qualcosa di più originale e innovativo. Invece, è venuto qui in Parlamento a rivendicare meriti di un Governo il cui bilancio è magro, di un Governo che aveva una forte investitura popolare e parlamentare e che oggi vivacchia in attesa della conversione di qualche deputato, un Governo frutto di una politica che ha espulso i moderati dal circuito delle decisioni, affidandole esclusivamente alle forze più estreme. Nel suo intervento, signor Presidente, non vi è traccia, neanche minima, di un'autocritica sulla diaspora dei moderati la cui unità lei ha rotto per un mero calcolo politico ed elettorale a vantaggio suo personale, di una parte di facinorosi di destra e della Lega Nord. Se oggi Casini, Fini, Rutelli, il Movimento per le Autonomie di Lombardo si trovano insieme in una nuova area della responsabilità è proprio perché lei ha scelto di non rappresentare più i moderati italiani, ma prevalentemente la destra populista che alimenta paure ed egoismi e che fa della demonizzazione dell'avversario la sua unica ragione di esistere. Per questo vogliamo che con le sue dimissioni si apra una fase nuova che porti alla formazione di un Governo che risolva i problemi delle famiglie e delle imprese italiane, un Governo che rimetta al centro della propria azione il Mezzogiorno d'Italia, un Governo che mantenga quello che promette e che promette solo ciò che può mantenere. Quello che lei guida, signor Presidente del Consiglio, è un Esecutivo che pretende di essere il Governo del fare, ma che si è rivelato il Governo del fare poco o, al massimo, del fare annunci; anzi, per l'esattezza, il Governo delle promesse mancate, prima di tutto per quanto riguarda la famiglia: niente quoziente familiare, niente *bonus* bebè, nessun sostegno alle giovani coppie, nessuna traccia della cedolare secca del 20 per cento sugli affitti. Ci troviamo nella situazione paradossale per cui, da un lato, si loda e si vanta l'attitudine delle famiglie al risparmio e si evidenzia come il debito delle famiglie italiane sia più basso di quello dei principali Paesi europei e, dall'altro, non si pongono le condizioni perché questa preziosa attitudine si consolidi e si rafforzi. Queste erano promesse su cui lei aveva chiesto prima il voto e poi la fiducia nel 2008 e queste sono promesse che lei e il suo Governo non avete mantenuto; promesse rinnovate ancora una volta lo scorso quando lei ha presentato un programma, l'ennesimo, che comprendeva giustizia, sicurezza, federalismo, Sud e fisco. Ma dov'è finita la riforma della giustizia? A fronte dell'urgenza di fare efficaci interventi legislativi autenticamente riformatori, annunciate un nuovo piano che prevede una riforma costituzionale che non potrà essere approvata in questa legislatura. Anche su sicurezza ed immigrazione il vostro bilancio è negativo se pensiamo ai mezzi e alle risorse che avete tagliato alle forze dell'ordine, qualcosa come due miliardi e mezzo di euro, o al *bluff* delle ronde. E che dire del fallimento della lotta all'immigrazione clandestina? Secondo gli ultimi dati disponibili, infatti, su oltre 52.000 clandestini fermati, solo 18.000 (il 34 per cento) sono stati effettivamente rimpatriati. È il dato più basso dal 1999 ad oggi. Tra i suoi cinque punti, signor Presidente, c'era anche il federalismo fiscale. I tanto decantati decreti attuativi del federalismo fiscale non dicono nulla; non c'è un numero, una cifra, una tabella. Siamo di fronte al federalismo delle chiacchiere che non responsabilizza ma divide; un federalismo che la propaganda leghista continua a spacciare come già realizzato quando fino ad oggi si è fatto poco o nulla e ciò che si è fatto non offre garanzie su quanto costerà all'Italia e su come funzionerà. Il suo, signor Presidente, è il Governo delle riforme finte, come quella dell'università; una riforma «a costo zero», anzi «a costo sotto zero», visto che la manovra economica ha stanziato un miliardo di euro per finanziarla mentre il ministro Tremonti gliene ha tagliato un miliardo e mezzo; una riforma che affida i suoi punti più qualificanti, come le disposizioni sulla qualità e l'efficienza del sistema universitario, a decreti attuativi per i quali dichiaratamente non ci sono risorse; una riforma che a tutto voler concedere entrerà in vigore fra dieci anni. Insomma, un'altra scatola vuota, come il federalismo, ed un'altra promessa mancata. Dei suoi cinque punti ho volutamente lasciato per ultimo il Sud. Il Sud che in questi due anni e mezzo è semplicemente sparito dall'agenda del Governo, con il taglio dei Fondi destinati alle aree sottoutilizzate o utilizzati a pioggia per scopi diversi. Ora lei ha ripreso a parlare di un presunto Piano per il Sud. Aspettiamo di vederlo; al momento si tratta solo di parole. Le do solo un dato per capire come non ci siamo e il dato riguarda le infrastrutture: solo il 39 per cento delle opere previste nel Piano infrastrutture strategiche è localizzato nel Mezzogiorno, e solo il 30 per cento delle delibere del CIPE riguarda opere per il Mezzogiorno. E questo la dice lunga sulle politiche meridionalistiche sue e dell'onorevole Bossi. l'Italia non cresce, non va avanti, non migliora, non funziona, non produce ricchezza. Ce lo dicono tutti, dal governatore della Banca d'Italia Draghi alla Commissione europea, da Confindustria al Fondo monetario internazionale, secondo il quale negli ultimi dieci anni l'unico Paese che è cresciuto meno di noi è Haiti. La crisi sociale che attraversa l'Italia è profonda; riguarda milioni di giovani disoccupati che non hanno alcuna speranza di entrare nel mondo del lavoro neanche da precari; riguarda le famiglie italiane che non riescono a pagare il mutuo di casa e non riescono ad assicurare un'istruzione dignitosa ai propri figli; riguarda le nostre imprese gravate da una tassazione eccessiva che li rende marginali nel quadro della competizione globale. È certo che nei prossimi mesi l'Italia sarà chiamata a scelte importanti per rendere stabile e strutturale il regolare andamento dei conti pubblici. Ma veramente, signor Presidente, lei ritiene che insieme a Bossi, soli come Thelma e Louise in quel bellissimo film del 1991 diretto da Ridley Scott, sarete nelle condizioni di affrontare senza una larga base politica e parlamentare i problemi difficili e complessi del Paese? Sappiamo tutti che lei non la pensa così e che, in realtà, insieme a Bossi ha un altro disegno in testa: quello di andare alle elezioni anticipate. Le elezioni anticipate sono la sua ultima fuga dalle realtà, utili a depistare gli elettori rispetto alle cose non fatte e alle promesse mancate. Servono a lei e servono a Bossi per raddoppiare il suo peso in Parlamento, soprattutto al Nord. Le elezioni anticipate, però, oltre che inutili e dannose, sarebbero la certificazione del suo fallimento che gli elettori punirebbero, oltre che un danno grave ed irreparabile all'interesse generale del Paese. Per questo, tra il suo governicchio e le elezioni anticipate, ci sono tante soluzioni migliori, a partire da un Governo di unità nazionale che faccia le riforme che faccia le riforme vere ed urgenti che servono all'Italia e che si formi con il concorso di tutti, innanzi tutto con il suo. Una volta tanto, signor Presidente, visto che tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile, compia un gesto di amore: si renda più utile che indispensabile, rassegnando le dimissioni. Il suo rifiuto di dimettersi non è un atto di coraggio ma di debolezza, che non fa onore a lei e non fa il bene del Paese. Proprio perché vogliamo il bene del Paese, anche questa volta le votiamo contro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, signore e signori Ministri,

Permane in molti lo stupore di fronte ad un'eclissi tanto rapida del sole sfolgorante della vittoria sulla sua Invincibile Armada. Ricordiamo tutti i numeri del voto di fiducia del 30 settembre scorso (che definirei una squisita vittoria di Pirro), così così celebrati dai suoi cantori come prova di esistenza in natura del gigante Anteo che, atterrato, dalla terra riceve nuovo e più grande vigore. Eppure, siamo a questo. Parafrasando «vedo le mura e gli archi

perché quadri, di uno, di due o di quattro voti la sua maggioranza alla Camera dei deputati. Se vuole vincere quello stupore (immagino, come è legittimo, che lei sia rabbioso), non basta evocare la categoria del tradimento: quella è buona per l'*epos*, ma non aiuta a capire. Per capire, agli umani sono normalmente richiesti un faticoso esercizio di umiltà, l'abbandono di un punto di vista che comincia e finisce in se stessi, e un poderoso senso della realtà. Noi, che siamo i suoi avversari, le diciamo le ragioni che abbiamo visto, sempre più velocemente, causare eventi imprevedibili per il suo Governo e per l'Italia. Ragioni che non sono l'atto di superbia di un arcangelo, cioè - per uscire dalla metafora - il tradimento del presidente Fini. La prima ragione sta in questa legge elettorale e, in particolare, proprio in quella norma sul premio di maggioranza che lei non intende in alcun modo cambiare. Le ha fatto ipervalutare il suo consenso elettorale, che era di un terzo dell'elettorato, anche perché gli elettori della Lega hanno votato - appunto - Lega, tracciando una croce su un simbolo che recava non il suo nome, ma quello di Umberto Bossi, a segnare una prudente autonomia che lei ha ben conosciuto nel 1996. Lei si è creduto più forte di quanto non fosse. Errore strategico, in guerra come in politica, che si è saldato ad un altro errore più grave, risalente: quello di non essere stato capace di onorare le aspettative che aveva suscitato. Ne ha scritto Galli della Loggia su un giornale normalmente molto generoso con lei, il "Corriere «C'era l'idea che quello che nasceva, nel quadro di un bipolarismo finalmente conquistato, doveva essere, sarebbe stata, una destra liberale adeguata ai tempi (quindi liberista ma con giudizio, per ma decisamente anticorporativa), pregna degli umori della società civile, ma dotata di senso delle istituzioni, capace di esprimere un'adeguata cultura e capacità di governo». «Berlusconi non è stato capace di dare vita a nulla di tutto questo (...) La grande scommessa berlusconiana è fallita». Peraltro, il senatore Pera ieri ha detto cose analoghe. un errore grave perché su quella aspettativa, che non ha onorato, lei aveva fondato due convincimenti illusori: quello di avere saldato un'alleanza stabile e finalizzata con soggetti importanti (come i ceti produttivi), radicando una stabile rappresentanza di interessi; di interessi; quello di non avere avversari nel campo della destra. Di fronte al fallimento di quella illusione operata dai suoi Governi, la pretesa alleanza è diventata, come era ovvio e naturale, una convenienza utilitaristica, pronta a cedere di fronte all'incapacità di adottare politiche addirittura necessarie, come avviene oggi nella crisi. dovrebbe dirle molto che il tavolo spontaneo di produttori e sindacato per un nuovo patto sociale non è stato né pensato né convocato né diretto da lei o dai suoi Ministri. Significa che oggi, quando ci sono in gioco interessi vitali per il Paese, si prescinde da questo Governo e si fa da soli. Il presidente Fini e il suo movimento la insidiano sul suo stesso terreno, la destra italiana, il nostro campo avversario, tanto per essere chiari. E Futuro e Libertà sta tentando di rappresentare una destra europea, moderna, liberale, rispettosa della Costituzione: ma appunto, una destra. Ora, che a qualche furbacchione torni utile dire che Fini si è spostato a sinistra, è roba buona per comizi di paese e per mancanza di argomenti. Temo che quello che trae in inganno qualcuno è il muoversi di Futuro e Libertà nell'ambito della Costituzione, del rispetto della democrazia: ossia, un atteggiamento consueto consueto per le destre europee, ma roba forte, lo capisco, per un partito che - per dirla con la soavità dell'onorevole Verdini - di tali questioni se ne frega. Insomma, è chiaro: la crisi è esplosa nella sua maggioranza. Lei ha messo in pericolo il suo Governo, in grave difficoltà l'Italia. Il suo essere *tycoon* è diventato una debolezza. Ha cacciato il cofondatore. Ha aperto il fuoco con ogni mezzo, anche il più sgradevole. Ne ha fatto una questione personale. Ha proclamato: o me o nessuno. come ha detto il senatore Zanda - non ha capito e saputo affrontare la qualità politica della crisi della sua maggioranza, le sue ragioni, i suoi argomenti, e ha impedito al suo partito, ai suoi dirigenti politici di intervenire: un partito che ha avuto tanto credito dagli italiani, il quale, se fosse stato normalmente responsabile, avrebbe dovuto invitarla alle dimissioni e sostituirla con un altro alla guida del Governo. Presidente, responsabilità nei confronti del Paese e non tradimento del popolo, anche perché ormai lo sanno tutti che lei non è stato eletto dal popolo. Questa è una Repubblica parlamentare. Lei è qui per ricevere o vedersi negata la fiducia dal Parlamento. Allora, altro che crisi al buio in cui le opposizioni cacciano il Paese! Lei ha cacciato l'Italia, il suo Governo e il suo partito in una crisi politica, rischiosa e incerta, che dura da mesi. Che fare adesso? Noi rispondiamo di noi. Siamo il secondo partito del Paese, di gran lunga il primo delle opposizioni. Tutti capiscono che, senza il Partito Democratico, non c'è possibilità di cambiamento in Italia. Abbiamo un solo dovere: quello di mettere responsabilmente la nostra forza al servizio dell'Italia. E questo gli italiani - mi creda - lo capiscono. Potete raccontarla come vi pare, ma il punto è questo. Mettiamo quietamente, colleghi, la nostra responsabilità al servizio del Paese, pronti a farlo in quello che riteniamo necessario - salva, ovviamente, ogni prerogativa del Capo dello Stato - in un Governo transitorio di responsabilità che aiuti l'Italia a resistere alla crisi e che produca una nuova legge elettorale, pronti alle elezioni se - sciaguratamente per gli italiani - a questo voi ci portaste. Abbiamo per farlo le nostre proposte (quelle che fate finta di non conoscere e che storpiate per la vostra propaganda), dirigenti politici ed eletti, partito e quel popolo appassionato e civile che avete visto sabato a Roma in piazza San Giovanni. Ne abbiamo la serietà e l'esperienza. Infine, presidente Berlusconi, voglio onorarla, o meglio voglio onorare le sue pirotecniche conclusioni di ieri con un modesto contributo di verità. Sulla ricostruzione in Abruzzo mi pregio di fornirle una nota che le eviti di irritare ancora di più le vittime del terremoto con le strane e balzane cose che ha detto ieri in quest'Aula. Sull'emergenza rifiuti in Campania, le auguro di non vincere il Comune di Napoli, altrimenti non saprà più su chi scaricare la responsabilità della vostra incapacità. In ultimo, quanto al debito pubblico da lei evocato, le fornisco la serie storica dal 1972 (sono dati Bankitalia).

con il quale, in dispregio della sentenza della Corte costituzionale, si permetteva alle sue televisioni di trasmettere sul territorio nazionale. È con queste considerazioni e con le molte, importanti, di merito, svolte dai miei colleghi che, a nome del Partito Democratico, negheremo la fiducia al suo Governo e la invitiamo, per il bene dell'Italia, alle dimissioni.

signor Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, l'Italia voleva, vuole e vorrà una competizione democratica bipolare, nella quale servono grandi partiti. Il Popolo della Libertà ha unito il popolo del centrodestra e ha vinto tutte le sfide elettorali che ha affrontato dalla sua nascita. Ha valorizzato nel Governo, accanto a chi ha una consolidata esperienza, una classe dirigente giovane che si è dimostrata all'altezza delle gravose responsabilità. Mentre c'è chi sceglie i linguaggi ambigui e dal sapore antico, voglio ricordare che la fonte principale di legittimazione in politica è quella popolare. Nel 2008 il centrodestra ha ottenuto 17 milioni e mezzo di voti contro i 15 milioni del centro sinistra. Solo quando viene diviso il fronte moderato si offrono delle *chance* alla sinistra, che peraltro le ha utilizzate male. Nella legislatura 1996-2001 si alternarono tre Governi con divisioni e lacerazioni. E D'Alema, per governare poco e male, dovette realizzare una vergognosa operazione di acquisizioni nel fronte parlamentare del centrodestra. Dividere, cari colleghi, il fronte moderato è un errore politico che va evitato. Il presidente Berlusconi in questo dibattito parlamentare e in numerose altre occasioni parlamentari e politiche ha aperto ad un patto di legislatura, al riconoscimento di una diversa articolazione della maggioranza, all'approfondimento delle tematiche economiche, che non possono tuttavia ignorare il quadro di riferimento europeo. aperto ad una legge elettorale che, comunque, non potrà rinunciare ai principi del bipolarismo e di una democrazia maggioritaria che favorisca la governabilità. Ma ha anche ricordato che prima vengono le riforme costituzionali: l'elezione diretta del Premier, la riduzione del numero dei parlamentari, la revisione del bicameralismo e il federalismo. Chi ha presentato mozioni di sfiducia sa solo dire dei no: le elezioni? Per carità! Creerebbero instabilità. Berlusconi si dimetta oppure - peggio ancora - lasci per sempre la scena politica, o ancora - la situazione è migliorata tra 72 ore lo facciamo tornare. Proposte ispirate alla ritualità della vecchia politica, di cui l'Italia non ne può più. *(Applausi Quali sono le proposte alternative, gli schieramenti che da questa sera potrebbero governare in alternativa il Paese? Quelli che hanno perso le elezioni? Si vorrebbe cancellare la volontà degli elettori, creando una situazione in contrasto con i principi della sovranità popolare sanciti dalla nostra Costituzione, dicendo falsità. Si è parlato di economia il commissario europeo all'economia, Rehn, è venuto in Parlamento giorni fa e ha detto che l'Italia ha saputo tenere sotto controllo difficili conti pubblici ed ha escluso manovre aggiuntive. chi abbia più ragione, se un autorevole commissario europeo o gli improvvisati economisti della sinistra italiana che quando hanno governato hanno prodotto solo guasti; e potremmo dimostrarlo con numeri e fatti. Il presidente Berlusconi ha auspicato una ricomposizione dell'area moderata che, se unita, potrà governare bene e a lungo, garantendo quelle riforme essenziali per l'Italia. Abbiamo riformato la pubblica amministrazione, abbiamo garantito il mondo del lavoro e le imprese; e consentitemi, in una giornata in cui alcuni minacciano nuove violenze, di solidarizzare con chi ha preferito il dialogo sociale allo scontro di classe, con Raffaele Bonanni, ancora una volta minacciato e intimidito

Abbiamo riformato e riformeremo scuola e università. Abbiamo affrontato i temi dell'immigrazione, contenendo il tasso di clandestini. Abbiamo affrontato i temi della sicurezza. Altri schieramenti non sarebbero in grado, né oggi né domani, di esprimere una spinta riformatrice quale la nostra. Anche sul fronte della legalità forte è stato il nostro impegno per combattere il crimine, contrastare le cosche, rafforzare il carcere duro. Abbiamo dovuto contrastare campagne menzognere basate su poco credibili pentiti, spesso esibiti anche nelle TV pubbliche,

Questa è la vergogna che denunceremo davanti al Paese e nel Parlamento! Noi la mafia l'abbiamo combattuta. Qualcun altro mise lo Stato in ginocchio davanti alla mafia!

Voi avete ironizzato quando il presidente Berlusconi venne a parlare della crisi della Georgia e rivendicò dei meriti, e alcuni ironizzarono anche in quest'Aula. Ebbene, Hillary Clinton, il 1° dicembre, ha affermato che Berlusconi ha garantito in Afghanistan un sostegno generoso e ha lavorato in Europa con il presidente Sarkozy per la stabilizzazione della Georgia. Ha poi aggiunto che non vi è amico migliore che ha sostenuto le Amministrazioni Bush, Clinton e Obama, così confermando

criticare oggi una Federazione russa che faticosamente cammina verso la democrazia, quando avete applaudito, nel passato, l'Unione Sovietica. Oggi questo Governo difende l'interesse energetico ed economico dell'Italia in maniera costruttiva e serena negli scambi

bisognava passare attraverso le società costituite dal Partito comunista, che incassavano una regolare tangente! È storia! Poi

signor Presidente, ribadendo che nel 2008 Berlusconi e lo schieramento di centrodestra, con la Lega Nord e il Popolo della Libertà uniti, ha vinto le elezioni. Dal 2008 al 2010 ha poi vinto elezioni provinciali, comunali, regionali, abbinando alla fiducia parlamentare una fiducia popolare,

opera all'insegna di quella sigla citata anche da Giuliano Ferrara: TTB, cioè tutto tranne Berlusconi. Gli italiani lo vogliono, il Parlamento gli concede la fiducia, ma per accontentare qualche vecchio stratega di una politica fallita, Berlusconi, chissà perché, dovrebbe dimettersi. Ma certamente

che siamo disponibili ad ampliare il programma del Governo, a rafforzare con idee e persone ulteriori questo Governo e non altri Governi. Ma le dimissioni, no! Sarebbero una contraddizione con tutto questo spirito costruttivo che anche oggi è stato espresso! Le dimissioni no, dopo che si è insinuato anche il peggio! Berlusconi è a palazzo Chigi perché gli elettori lo hanno collocato lì e il Parlamento gli ha rinnovato la fiducia, non per oscuri motivi. la strada per rafforzare il Governo non è certo quella delle lacerazioni. Cerchiamo di ripartire insieme. Se facessimo scelte diverse, cari colleghi, metteremmo in discussione quanto di storico abbiamo fatto insieme: dare lo scettro al popolo e non agli apparati dei partiti. Questo è stato il cammino che abbiamo fatto insieme dal 1994 ad oggi. Quindi,

signor Presidente del Consiglio, colleghi, intervengo a nome della Südtiroler Volkspartei e anche a nome dei miei colleghi Pinzger e Peterlini. Il 30 settembre scorso, in occasione delle votazioni sulla questione di fiducia, nella nostra dichiarazione di voto abbiamo indicato chiaramente la posizione del nostro partito. La Südtiroler Volkspartei ha fatto una precisa scelta politica fin dall'inizio di questa legislatura: rimanere indipendenti senza patti o alleanze politiche a livello nazionale. Seguiamo quindi la politica dell'autonomia decisionale: guardiamo i fatti concreti e valutiamo nel merito i singoli provvedimenti. Noi della Südtiroler Volkspartei, pur avendo alcune riserve sull'operato del Governo, riteniamo sia un atto irresponsabile aver determinato questa crisi in un momento di particolare difficoltà economica sia del Paese che del contesto internazionale. Chi per problemi personali o di partito ha determinato la crisi deve assumersi la responsabilità di fronte al Paese! Questi problemi andrebbero risolti in seno alla maggioranza stessa, mantenendo il doveroso distacco dai ruoli nelle istituzioni rivestiti dai protagonisti LNP)*:sarebbe opportuno mantenere da queste lontane le posizioni delle rispettive cariche politiche. *(Applausi Signor Presidente, ci auguriamo che questa crisi venga finalmente superata: non possiamo perdere altro tempo, i cittadini ci hanno dato l'incarico di lavorare per loro e per il bene del Paese. Per senso di responsabilità e per tenere fede alla nostra linea politica, ossia di operare in autonomia decisionale, annuncio la nostra astensione che, nel rispetto del Regolamento del Senato, si traduce in una non partecipazione al voto.

Non ero stata preannunziata perché io amo ragionare con me stessa e con la mia coscienza. Anch'io sono stata eletta nella lista «Il Popolo della Libertà», ma non sono entrata nel partito «Il Popolo della Libertà»,

politico: una nicchia del mio interesse per il Mezzogiorno d'Italia. Vede, Presidente, mi è molto dispiaciuto che lei non abbia sottolineato di più il suo interesse per il Mezzogiorno. È una battaglia nella quale ho creduto e crederò fino in fondo, comunque vadano le cose, sia che lei decida di far andare il Paese ad elezioni anticipate, sia che lei decida di voler pensare ad una maggioranza sostanzialmente più coesa e qualitativamente anche più interessante e con degli obiettivi che siano molto più precisi e pregnanti di quelli che invece sono stati indicati fino a questo momento. Presidente, sinceramente non credo che quel piano per il Sud, così come è stato presentato, sia realmente denso di contenuti. Non so con chi, quando, come, con quali finanze, e se veramente lei lo vorrà portare avanti, ma non mi voglio aggiungere alla schiera di coloro che si sono divertiti in questo periodo a fare una sorta di tiro alla fune. Non mi piace, soprattutto come cittadina italiana, che in Italia ci sia un Governo che non riesce a governare veramente e che deve chiedere continuamente la fiducia al Parlamento. Credo che lei la fiducia l'abbia avuta a suo tempo dagli italiani, come ho provato a dire in poche parole ieri. Tra l'altro, non credo che lei si sia addormentato mentre stavo parlando, come qualcuno ha scritto sui giornali. Anzi ho visto che lei ha ascoltato tutti con grande attenzione e di questo gliene siamo grati.

coloro i quali sono contrari risponderanno no; coloro i quali intendono astenersi risponderanno di conseguenza. Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio la chiama.